Risponderò congiuntamente ai senatori Gramazio e Tofani in merito alla loro richiesta di conoscere le iniziative che il Governo intende adottare per affrontare i problemi derivanti della presenza di numerosi Rom nella città di Roma e nel Lazio. questioni che hanno posto sono di tale rilievo che nei patti per la sicurezza, siglati dal Ministero dell'interno con i sindaci delle grandi aree metropolitane, vi è un apposito capitolo dedicato alla presenza delle popolazioni Rom. I problemi specifici per la presenza di comunità Rom a Roma, nella quale risultano presenti circa 4.900 persone di varia nazionalità, dislocate nei 24 campi autorizzati, sono stati portati più volte all'attenzione del Ministero dell'interno che ha sensibilizzato il prefetto perché individuasse proposte sia relativamente alla tutela dei campi più a rischio, sia per la delocalizzazione, con il coinvolgimento della regione Lazio, in altre realtà territoriali. Proprio in merito a ciò, ci sono state numerose riunioni con i soggetti istituzionali coinvolti, anche se debbo dire che gli esiti non sono stati positivi a causa delle preoccupazioni e dell'opposizione dei sindaci. È questo anche il caso dell'area individuata nel comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano, in provincia di Frosinone, cui fa riferimento il senatore Tofani nella sua interrogazione. Presso la prefettura di Roma opera un gruppo di lavoro per il controllo, lo sgombero e la messa in sicurezza dei campi Rom abusivi. Sono stati chiusi i campi di Tor Pagnotta e la parte abusiva di Villa Traili, inoltre, sono state sgomberate alcune baraccopoli abusive, tra le quali quella sorta nell'area di Tor Vergata, e sono calendarizzati altri interventi di bonifica. La massima attenzione verrà posta affinché i campi smantellati non vengano ricostituiti. A partire dal 18 maggio è operativo il "patto per Roma sicura", sottoscritto alla presenza del ministro Amato. Nel patto è previsto che viene costituita dal Prefetto, d'intesa con il Sindaco, presso la Prefettura di Roma, una commissione intesa a promuovere interventi risolutivi delle esigenze di contenimento delle popolazioni senza territorio, nonché inclusione sociale, attraverso, rispettivamente: la costruzione di quattro villaggi della solidarietà in aree attrezzate in grado di ospitare circa mille persone - ciascuno da realizzare su aree comunali o demaniali disciplinati da specifici regolamenti di gestione; programmi di abbattimento di insediamenti abusivi, con successiva riqualificazione delle aree liberate. Dell'esito dei lavori della commissione sarà informata la Regione Lazio. Ai fini delle iniziative di cui sopra - utili anche per la prevenzione di possibili occasioni di tensioni sociali - la Commissione provvederà ad individuare, entro nove mesi, i predetti villaggi; tali strutture verranno gestite dal Comune stesso, fruendo di servizi di mirata vigilanza effettuata dalle forze di polizia, nell'ambito delle proprie competenze funzionali e del rinforzato dispositivo di controllo del territorio. Le forze di polizia provvederanno nel contempo ad intensificare l'attività di vigilanza dedicata sugli attuali insediamenti autorizzati. Nei confronti degli insediamenti abusivi, ovvero di eventuali situazioni di pericolo accertate in quelli autorizzati, la commissione definisce un programma di prevenzione e di recupero delle situazioni di illegalità e di degrado, nell'ambito del quale potranno essere, ove necessario, assicurati servizi di controllo integrati, disposti dalle autorità di pubblica sicurezza, secondo le specifiche attribuzioni, e supportati da collaterali servizi comunali. Per esigenze di vigilanza e di intervento di cui sopra viene disposta l'assegnazione di ulteriori 150 elementi (75 della Polizia di Stato e 75 dell'Arma dei carabinieri). Relativamente alla situazione del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano, è noto che la decisione cui fa riferimento il senatore Tofani è stata revocata. Concludo ricordando che nella legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), nell'articolo 1, commi 1267 e 1268, è stato istituito il Fondo per l'inclusione sociale degli immigrati al fine di favorire l'inclusione sociale dei migranti e dei loro familiari. Al momento sono in preparazione gli atti e i provvedimenti concernenti l'utilizzazione del fondo da parte del Ministero della solidarietà sociale, di concerto con il Ministero per i diritti e le pari opportunità; nell'ambito delle priorità di intervento che riguardano marginalità sociale,

La ringrazio, signora Sottosegretario, per la ufficializzazione, anche in questa sede, del fatto che sia stata revocata quella decisione; quindi, ne prendo atto con soddisfazione. Desidererei sapere, se possibile, e lo chiedo anche nell'interrogazione, atteso che il sindaco del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano è stato direttamente convocato dal prefetto di Roma, in qualche modo bypassando il prefetto di Frosinone, quale procedura si è seguita, cioè che natura giuridica e che rapporto c'è tra il Ministro, il prefetto di Roma, il prefetto di Frosinone e il sindaco del Comune di Sant'Ambrogio sul Garigliano. Desidero, altresì, aggiungere un dato importante: quando si individuano queste aree, credo non si possa non considerare anche la destinazione delle stesse; lo dico perché lei ha svolto un intervento più ampio sul tema, è anche comprensibile, visto l'argomento. Ebbene, nello scegliere le aree, diventa preoccupante immaginare che si vada ad individuare un'area attrezzata e destinata a campeggio in una zona in cui è necessario lo sviluppo del turismo, atteso che stiamo parlando dei Comuni della «*terra Sancti Benedicti»*. Quindi, auspico che, nelle scelte congiunte, tra Regione, Ministero dell'interno, prefetto di Roma o chi per loro, non si metta il dito su un punto particolare della carta geografica e si dica: qui può andare bene.

per l'interno. Quando è stato lanciato l'allarme e tutti i quotidiani romani e nazionali hanno parlato di alcuni problemi che riguardavano l'aumento della presenza dei nomadi nella nostra città, la giornalista Coletti, su «Il Tempo», riportò frasi precise del prefetto di Roma. Orbene, riallacciandomi a quanto diceva poc'anzi il collega Tofani, vogliamo capire se le competenze del prefetto di Roma riguardano l'intero territorio regionale

Quindi, come si interviene e quali iniziative intende prendere il Ministero a garanzia dell'ordine e della sicurezza? Non devo certo dire a lei, che è persona attentissima a questi problemi, che alcuni giorni fa in due campi nomadi attrezzati della città di Roma, durante una perquisizione dei Carabinieri, è stata ritrovata un'ingente quantità di droga che doveva essere smerciata e i capi vivevano in quei

numerosa refurtiva di appartamenti svaligiati nella città di Roma. Quindi, si auspica maggiore attenzione in tal senso e di sapere, come ha detto il collega Tofani, se il prefetto di Roma è stato investito di una superprefettura del Lazio.

molto contenta dell'interlocuzione che si può sviluppare con serenità su una questione molto complessa. Quindi, credo sia davvero importante che anche il confronto, pur muovendo da posizioni e valutazioni diverse,

particolare allo stesso senatore Gramazio, firmatario di questa interrogazione, che riguarda specificamente il fenomeno dell'accattonaggio e della mendicità; mendicità; fenomeno che spesso rappresenta il drammatico esito che finisce per accomunare una pluralità di situazioni individuali e di percorsi di marginalità e di esclusione sociale anche molto diversi gli uni dagli altri. Occorre, in ragione di ciò, evitare di incorrere in eccessi di semplificazione o generalizzazione, in quanto la molteplicità delle cause remote di queste manifestazioni di povertà e di sofferenza rende più difficile l'approccio unitario ad una problematica che, del resto, non può essere affrontata e contrastata solo con interventi di pubblica sicurezza, ma al contrario richiede il più delle volte interventi qualificati di carattere sociale ed assistenziale. Il fenomeno, presente a Roma così come nella generalità delle grandi città, in questa realtà ha registrato un incremento già a partire dai primi anni Novanta, in coincidenza con la disgregazione dell'ex Jugoslavia e la diaspora dai Balcani, dai quali provengono molti dei Rom tuttora presenti nell'area metropolitana.

Nella sua forma criminale più odiosa e ricorrente, lo sfruttamento dell'accattonaggio minorile, il fenomeno della mendicità ai semafori, è da tempo noto alle autorità, che per contrastarlo operano anzitutto sotto il profilo preventivo, ad esempio attraverso azioni per la riduzione della dispersione e dell'abbandono scolastico, per il sostegno alla genitorialità difficile,

se non seguiti nel loro percorso sul nostro territorio, spesso finiscono arruolati nelle fila delle criminalità che li sfrutta. Anzi, le nostre Forze di polizia ci dicono che alcuni minori partono dal

Accanto a queste azioni preventive vi sono interventi sotto il profilo repressivo, con mirate, specifiche operazioni di polizia volte ad individuare e perseguire penalmente i responsabili dello sfruttamento. Su questo tema a Roma c'è una particolare sensibilità, che si estrinseca anche in specifiche attività realizzate dall'ente locale e dalle organizzazioni del terzo settore; penso, ad esempio, al Centro diurno per il contrasto alla mendicità infantile promosso dal Comune, con la partecipazione di una vasta platea di soggetti pubblici e privati. Relativamente meno noto e ricorrente, ma non per questo meno grave ed odioso, è il fenomeno cui fa riferimento l'articolo de «Il Tempo» citato dal senatore Gramazio, cioè quello dello sfruttamento organizzato della mendicità degli adulti, tema ancora oggi sui quotidiani. Per lo più, si tratta di invalidi e mutilati provenienti dai Paesi dell'Est. È anche questa una problematica inerente allo sfruttamento e alla riduzione in schiavitù di persone ed è all'attenzione delle Forze di polizia, che vi stanno dedicando specifiche attività di vigilanza e di indagine.

preciso che, secondo quanto riferito dalla questura di Roma, risulta che, a seguito dei frequenti servizi di controllo effettuati nella zona dalle Forze di polizia, non si sono più riscontrate manifestazioni del fenomeno.

di un accattonaggio particolare: si attendeva la disposizione e l'ordine, poi si usciva e ci si metteva al semaforo. Credo che la denuncia del quotidiano romano il mio intervento nei riguardi del prefetto e del questore siano valsi poi un intervento di polizia in questo senso. Sono convinto della sua risposta, giustissima,

un'attenzione maggiore da parte delle autorità. Il Comune di Roma ha un nucleo di polizia municipale organizzato per questo, ma la città di Roma è vasta e il nucleo è piccolo; però, quando vi sono queste segnalazioni da parte del Ministero dell'interno dovrebbe esserci un richiamo agli organi di polizia affinché, quando si riscontrano queste situazioni, si intervenga o direttamente o con la segnalazione nei riguardi dell'apposito nucleo del Comune di Roma, per tentare di arginarle ed evitare situazioni

in sotterraneo avviene con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Regione interessata dalla realizzazione dell'impianto. L'assolvimento delle relative procedure rientra nelle competenze del Ministero dello sviluppo economico in base, principalmente, alla legge 17 gennaio 1974, n. 170 n. 170 (modificata dal decreto legislativo n. 164 del 2000) e alla legge 23 agosto 2004, n. 239, nonché al decreto del Ministro delle attività produttive 26 agosto 2005, recante norme sulle "Modalità di conferimento della concessione di stoccaggio di gas naturale in sotterraneo, approvazione del relativo disciplinare tipo nel quale sono previste le modalità di attuazione delle attività di stoccaggio, gli obiettivi qualitativi, i poteri di verifica, le conseguenze di eventuali inadempimenti". In particolare, il decreto legislativo n. 164 del 2000 ha introdotto, per la prima volta in Italia, la possibilità di stoccare gas naturale in unità geologiche profonde, compresi gli acquiferi salini profondi, in analogia con quanto già fatto in altri Paesi, quali Stati Uniti, Canada, Francia, Germania, Danimarca e Russia. A seguito della domanda presentata dalla Indipendent Gas Management (IGM), nel luglio 2002, è stato pubblicato sul numero di agosto dello stesso anno del "Bollettino ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia", presente sul sito Internet del Ministero, la comunicazione rivolta agli operatori del settore sulle istanze "Rivara Stoccaggio", in provincia di Modena, e "Canton Stoccaggio", in provincia di Venezia, con l'indicazione delle aree nell'ambito delle quali la società istante avrebbe potuto realizzare gli impianti per la movimentazione del gas naturale da stoccare in idonee formazioni geologiche presenti nella profondità del sottosuolo. Sulla base dell'esame degli allegati tecnici presentati dalla IGM, nonché dei dati a conoscenza dei competenti uffici del Ministero, sono state eseguite sulle due istanze apposite istruttorie e redatte specifiche relazioni portate all'attenzione del comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, organo consultivo del Ministero sulle problematiche attinenti la ricerca, la coltivazione e lo stoccaggio in sotterraneo degli idrocarburi, nel luglio 2004. Nella seduta del 15 luglio 2004, il comitato tecnico, formato da esperti del settore appartenenti al mondo accademico, da funzionari delle amministrazioni interessate, fra le quali il Ministero dell' ambiente e le Regioni di volta in volta interessate, ha esaminato le relazioni predisposte dai competenti uffici del Ministero dello sviluppo economico, in relazione alla fattibilità geologica e mineraria del progetto, esprimendo parere favorevole al progetto di Rivara. Lo stesso comitato tecnico, nella medesima riunione, ha ritenuto opportuno rinviare l'esame del progetto relativo a Canton al momento successivo ad un eventuale esito favorevole della fase di accertamento del progetto Rivara, in quanto la formazione geologica presente nel sottosuolo veneto risultava più superficiale di quella di Rivara. Il 12 luglio 2005, la società istante è stata invitata a chiedere al Ministero dell'ambiente l'avvio del procedimento di *screening* ambientale per il progetto Rivara, al fine di verificare la necessità o meno di una valutazione di impatto ambientale ai sensi della vigente normativa. La IGM ha, comunque, deciso di sottoporre direttamente il progetto a VIA e il 15 settembre 2006 ha pubblicato l'avviso sui quotidiani nazionali e locali per l'inizio del relativo procedimento. In merito alle specifiche richieste avanzate nell'atto in esame, oltre ad evidenziare che finora non è stata conferita alcuna autorizzazione o concessione, si precisa che sono tuttora in corso, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, le valutazioni tecniche inerenti gli impatti ambientali. Nel caso di esito favorevole della procedura di VIA, il processo di valutazione e decisione circa la realizzazione del progetto di dettaglio verrà ripreso da questo Ministero, come previsto dalle norme vigenti, con lo strumento della conferenza dei servizi disposta dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e, quindi, con il completo coinvolgimento delle istituzioni locali e degli organismi tecnici competenti alla realizzazione del progetto; ciò al fine di approvarne le caratteristiche definitive, dichiararne la pubblica utilità, procedere alle varianti urbanistiche, apporre il vincolo per gli eventuali espropri dei terreni e, quindi, solo allora, conferire la concessione di stoccaggio, di concerto con il Ministero dell' ambiente e d'intesa con la Regione. Si precisa, inoltre, che la società IGM, a tutti gli effetti da ritenersi istante e non concessionaria, ha presentato una documentazione inerente l'esperienza e le conoscenze specialistiche dei mercati energetici in via di liberalizzazione vantate dai soci, accompagnata dall'atto costitutivo della società a responsabilità limitata e dal certificato di iscrizione alla camera di commercio di Livorno, nonché da una nota di credito certificata da una banca statunitense d'importo ritenuto idoneo a garantire l'attività preliminare di progettazione finalizzata al compimento dell'*iter* procedurale per il conferimento della concessione. Si sottolinea, altresì, che nel corso della procedura è stata acquisita agli atti una nota rilasciata da rilevante operatore europeo del mercato del gas naturale su un accordo di confidenzialità sottoscritto con la IGM relativo al progetto di stoccaggio di Rivara. Infine, si precisa che non essendo stata rilasciata alcuna concessione, allo stato attuale non risultano depositate fideiussioni o prestazioni di altre garanzie, non richieste in questa fase procedurale del conferimento. Quanto alla richiesta relativa alla necessità che la IGM «integri la relazione per gli aspetti riguardanti la geochimica e la sismicità delle aree interessate», si precisa che tali aspetti, indubbiamente fondamentali, sono stati trattati nell'ambito della procedura di valutazione d'impatto ambientale, realizzata presso il competente Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Al riguardo, tale Ministero ha fatto presente che, in sede di istruttoria tecnica, la Commissione preposta alla procedura di ha richiesto significativi elementi integrativi, rispetto alla documentazione già prodotta, che deve essere presentata a tutte le Amministrazioni che concorrono alla procedura medesima, proprio in questi giorni.

soprattutto per un'altra serie di vicende che abbiamo riportato anche nell'interrogazione, che ci fosse stata una costituzione *ad hoc* soltanto per presentare la società. proprio per l'effetto del cosiddetto decreto Letta che lei citava, signor Sottosegretario, dove si parlava giustamente della separazione delle attività di trasporto, vendita e stoccaggio del gas,

utilità solo per i soggetti che operano nella commercializzazione del gas. Lei, signor Sottosegretario, ci dice che, ovviamente, non essendo ancora società concessionaria, per fortuna, non sono state depositate le fideiussioni, ma

Sappiamo che la VIA è in corso e allora ci preme sottolineare anche che vi è una fortissima preoccupazione nel territorio (che lei conosce benissimo), tant'è che la provincia di Modena e l'unione

in cui si è potuto intervenire in sicurezza perché si trattava di aree scarsamente popolate. Chiedo, quindi, anche la disponibilità al Ministero dello sviluppo economico di considerare questo progetto con particolare attenzione, proprio per la delicatezza della proposta. **Saluto

Signor Presidente, in risposta all'interrogazione presentata dal senatore Possa, si osserva che la maggior parte del mondo scientifico internazionale da tempo ritiene che le attività antropogeniche, svolte dal periodo *post*-industriale ad oggi, rappresentano la principale causa del surriscaldamento del pianeta. Tale conclusione è stata ribadita nel quarto rapporto di valutazione, approvato dal gruppo di lavoro n. 1 lo scorso febbraio, al quale fa riferimento anche il Ministero dell'ambiente. Al riguardo, occorre evidenziare che l'IPCC è un organismo delle Nazioni Unite, istituito nel 1988 dalla Organizzazione mondiale per la meteorologia e dal Programma ambientale delle Nazioni Unite, allo scopo di fornire a chi fa politica una valutazione obiettiva e corretta della letteratura tecnico-scentifica e socio-economica disponibile in materia dei cambiamenti climatici, impatti, adattamento e mitigazione. Per quanto concerne, in particolare, il fenomeno dell'incremento della temperatura media globale, si evidenzia che l'IPCC ha calcolato tale incremento considerando una media tra le temperature rilevate sulla superficie terrestre e quelle rilevate sulla superficie marina, tenendo presente, altresì, l'impatto delle "isole di calore" urbane, certamente reale, ma di entità talmente limitata da essere stimato in 0,006 gradi centigradi per decennio. Per quanto attiene, invece, il tema specifico delle responsabilità del riscaldamento globale in atto, si fa presente che nelle conclusioni contenute nel documento "Sintesi per i decisori" predisposto dal gruppo di lavoro n. 1 del quarto rapporto di valutazione dell'IPCC, si rileva che "la maggior parte degli aumenti nella media delle temperature globali dalla metà del XX secolo è, molto probabilmente, dovuta all'aumento osservato della concentrazione di gas ad effetto serra causato dall'attività umana". La scelta collegata all'obiettivo di contenere l'aumento della temperatura media globale del pianeta entro i 2 gradi centigradi, al fine di limitare gli impatti sulla società e sui sistemi naturali, dipende, comunque, da considerazioni soggettive sull'entità del rischio ammissibile. A tal riguardo, la "Sintesi per i decisori" predisposta dal gruppo di lavoro n. 2 del quarto rapporto di valutazione dell'IPCC, approvata nell'aprile scorso, ribadisce

per la biodiversità e per i beni e servizi che essa fornisce, come l'acqua e il cibo". Infine, è opportuno rilevare che, già prima della pubblicazione del citato rapporto di valutazione, in sede di Consiglio europeo svoltosi nella primavera 2005, i Capi di Stato e di Governo dell'Unione Europea avevano affermato che "per realizzare l'obiettivo ultimo della Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, l'aumento mondiale annuo della temperatura di superficie non deve superare di 2 gradi centigradi i livelli preindustriali"; pertanto, non appare congruo intraprendere iniziative presso la Commissione europea per rivedere gli obiettivi già stabiliti. L'obiettivo di limitare l'incremento della temperatura globale a non più di 2 gradi centigradi corrisponde, infatti, a valutazioni condivise dalla stragrande maggioranza della comunità scientifica, alle quali il nostro Paese - insieme a tutti i suoi *partner* europei -si è sempre ispirato anche nel recente passato.

il primo, con 1,66 watt al metro quadro, è costituito dall'anidride carbonica da combustibili fossili, ma poi c'è, ad esempio, il metano dovuto all'agricoltura, ben 0,48 watt al metro quadro;

"Il link apre una nuova finestra") riguardante il Servizio dell'emergenza sanitaria nel Lazio. Ieri, con una delibera della Giunta regionale, sono stati tagliati 14 milioni di euro al Servizio dell'emergenza sanitaria. Da quest'oggi i sindacalisti della CGIL, CISL, UIL, dei sindacati autonomi sono a manifestare sotto la Giunta regionale del Lazio per tentare di comprendere per quale motivo nell'accordo Stato-Regione sono stati tagliati fondi all'emergenza sanitaria. Non devo ricordare a lei, gentile Presidente, che è attento conoscitore dei problemi di questa Regione, che l'ARES 118 è il miglior servizio di emergenza sanitaria d'Italia e che dispone del miglior servizio di eliambulanza, per cui la Protezione civile e il Ministero degli interni fanno ad esso riferimento ogni volta che vi è un'emergenza in ogni parte d'Italia. Il taglio di 14 milioni di euro, come denuncia il presidente della Commissione sanità della regione Lazio Dalia, che attacca direttamente